I problemi che possono derivarne al nostro Paese li possiamo immaginare: abbiamo rapporti economici, di lavoro, turistici.

talché il mistero venisse risolto. Adesso i colleghi della passata opposizione, oggi maggioranza, non lo fanno più. Mi viene da pensare, quindi, che non fosse una giusta motivazione quella per cui prendevano la parola, ma piuttosto un atteggiameno dilatorio. Non fate oggi quello che facevate ieri e rifate quello che

ringrazio, senatore Ferrara, per averci ricordato questa ricorrenza, anche perché personalmente, ma credo di interpretare il pensiero di molti, ogni volta che ricorre questa data mi vergogno come politico e come uomo.

in quanto esso intende estrapolare i lavoratori autonomi da quanto disposto

Né può soccorrere il riferimento alla raccomandazione 2003/134 del Consiglio europeo del 18 febbraio 2003,

2, lettera *c)*. Ricordo che, per quanto riguarda i lavoratori autonomi, appare più opportuno procedere nei termini già convenuti con le associazioni di categoria, ovvero limitatamente ai dispositivi di protezione individuale e al controllo sanitario periodico. Queste sarebbero già novità significative rispetto all'ordinamento vigente, che non prevede alcun coinvolgimento dei lavoratori autonomi nelle discipline relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

soprattutto di certe categorie ed in certe tipologie di lavoro, rivestono una loro specificità, che non può essere inserita in una legge o in un provvedimento generale che, invece, riguarda le imprese nel vero senso del termine. Pertanto, pensare di ampliare tutta una serie di obblighi

Signor Presidente, vorrei motivare l'orientamento favorevole del Gruppo di Forza Italia all'emendamento 1.17 del senatore Poli, laddove segnala la necessità di articolare la disciplina: «per specifiche tipologie di «per specifiche tipologie di lavoro, settori di attività o età dei soggetti». Sembra, questa, un'articolazione più congrua rispetto a quella del testo all'esame.

giungiamo alla disposizione cui mi sono più volte richiamato, quella già prevista dalla bozza di testo unico che è stata portata all'esame

relativa alla sicurezza per quanto riguarda i lavoratori autonomi. Non comprendo la ragione dell'opposizione del Governo a questa specificazione relativa all'introduzione di una nuova regolazione per quanto riguarda i lavoratori autonomi. Infatti, la materia è stata lungamente negoziata con le parti sociali

che riteniamo giusta la posizione verso l'imprenditore che si rende colpevole rispetto alla normativa nella delicata materia della tutela del lavoro;

chiediamo il dimezzamento, ossia una pena giusta e severa, ma non tale da impedire all'azienda di sopravvivere, specialmente in questi settori di microimprenditorialità, come alcuni dell'agricoltura.

siamo entrati nel punto forse più delicato del provvedimento. per mia disattenzione, i precedenti due emendamenti sono stati votati senza una opportuna attenzione da parte dell'Aula. 1.702, presentato dal senatore De Poli, riprende lo stesso tema che tornerà poi in molti emendamenti successivi. Il Governo propone un apparato sanzionatorio che non appare funzionale a creare una adeguata deterrenza rispetto ai comportamenti in violazione delle delle disposizioni che pure il testo unico vorrà meglio organizzare. Si dice, in particolare, da parte del senatore De Poli, che la delega per la riorganizzazione dell'apparato sanzionatorio «deve rispondere ai criteri di coerenza, proporzionalità, rischiosità». Non vedo come si possano negare questi criteri elementari, anche se, invero, molte delle disposizioni che poi esamineremo non appaiono proprio coerenti, proporzionali e caratterizzate da attenzione soprattutto alla dimensione del rischio. Credo quindi opportuno adottare un principio di esercizio della delega di questo tipo per regolare in conseguenza tutta la disciplina sanzionatoria.

ritorna il tema dell'alternatività tra arresto e ammenda. Nell'ordinamento attuale, arresto e ammenda sono sempre sanzioni disposte in alternativa tra di loro, nel senso che è possibile evitare l'arresto attraverso il ravvedimento operoso, che consiste nella rimozione dei fattori che possono determinare un danno per il lavoratore

che sembrano tra di loro contraddittori, perché da un lato si afferma la volontà di incoraggiare il ravvedimento operoso, mentre, dall'altro, si prevede la possibilità della sanzione dell'arresto senza l'alternativa dell'ammenda, quindi senza la possibilità di evitare l'arresto con comportamenti che costituiscano ravvedimento operoso.

sulla base di una delega. Il Senato, il Parlamento nel suo insieme, sta abdicando ad una funzione legislativa che la Costituzione gli assegna non su dettagli tecnici che potrebbero avere senso in una disciplina del genere, su dettagli che riguardano - che so - le attrezzature, il particolare materiale da usare, che sarebbe troppo lungo forse dibattere in quest'Aula, ma su arresto e su ammende molto pesanti. Stiamo veramente ponendo in essere una una privazione, un'abdicazione - lo ripeto - del Senato rispetto alla funzione che gli è propria e che gli è affidata dalla Costituzione. Nel merito, ci stiamo ci stiamo affidando a questo Governo per stabilire tutta una vasta articolazione di sanzioni,

sul lavoro, introdotto con il maxiemendamento alla finanziaria. Credo che non possiamo accettare una cosa di questo genere e ricordo - se ci fosse qualche dubbio sulla possibilità di legiferare in questa materia

laddove si dispone «l'applicazione ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, delle disposizioni sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche». Vorrei ricordare che la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, che può condurre fino all'interdizione dall'esercizio di attività di amministrazione di società, di società, nell'ordinamento attuale si connette a reati di carattere doloso. Per la prima volta, invece, si introdurrebbe una responsabilità per reati di omicidio colposo e lesioni colpose. Oltretutto, l'interdizione degli amministratori produrrà ragionevolmente una difficoltà nella continuità dell'attività aziendale con danno per terzi incolpevoli, come sono i lavoratori. manifesta sproporzione tra la sanzione e l'obiettivo che essa si prefigge; si determina una instabilità non giustificata nella vita dell'impresa e nella condizione dei lavoratori.

doveroso circoscrivere la responsabilità.

propria della 5a Commissione in ordine ai problemi conseguenti alla doverosa applicazione dell'articolo 81 della Costituzione. Questo, quindi, ci ha dovuto trovare

per poter formulare i propri bilanci in modo conseguente alla utilizzazione delle rinvenienze delle sanzioni pecuniarie per i reati di cui alle lettere precedenti e la utilizzazione per una

di destinare gli introiti delle sanzioni pecuniarie "per interventi mirati alla prevenzione, a campagne di informazione e alle attività dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende unità sanitarie locali". Mi sembra un orientamento di tutto interesse.

e facciamo oggettivamente fatica a capire perché ci sia questo invito al ritiro, alla sua trasformazione in ordine del giorno e quant'altro. Proprio dal punto di vista economico non capisco quale possa essere il problema per la 5a Commissione,

complesso. Abbiamo anche qui evidenziato in tutte le discussioni dei giorni scorsi che uno dei problemi più importanti della questione sicurezza è proprio la diffusione della cultura della sicurezza, la diffusione della consapevolezza dei rischi che si corrono nei posti di lavoro, che spesso sono sottovalutati, tant'è che la maggior parte o comunque moltissimi incidenti avvengono proprio per disattenzione o per eccesso di sicurezza da parte

avanzino poi dei fondi che vengono destinati a tutt'altre questioni, magari anche giuste, ad esempio l'edilizia scolastica, universitaria, eccetera, che possono essere certamente nell'interesse del Paese ma non certo nell'interesse dell'istituto specifico. Abbiamo invece una quantità notevole di aziende esempio, hanno già problemi di bilancio, di costo del lavoro e tutto ciò che ne consegue, e che pagano premi che ormai, per quanto riguarda le imprese artigiane e le imprese piccole e medie sono di due-tre volte superiori alle uscite per copertura di infortuni della stessa categoria di aziende.

Presidente, mi scusi, ma su questo emendamento c'era il parere contrario della Commissione bilancio.

rispetto agli organici degli organismi di vigilanza in relazione alle condizioni ambientali, alle concentrazioni di lavoratori e alle tipologie di lavori, poiché mi pare che la distribuzione degli organici di vigilanza debba essere rapportata a tali elementi.

svolgo questa dichiarazione di voto soprattutto per richiamare l'attenzione della maggioranza e, in particolare, quella dei componenti della 12a Commissione, perché perché questo emendamento altro non è che un adeguamento al parere espresso dalla nostra Commissione in maniera unanime e così ben descritto dal senatore Silvestri. Voglio ricordare che quanto previsto alla lettera *g)* del comma 2 rischia di portare una sequela di polemiche. Infatti le due figure professionali in oggetto sono state già normate recentemente con il decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che individua le capacità e i requisiti professionali richiesti agli addetti e ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori,

approvata a larghissima maggioranza in quest'Aula per rispondere ad una oggettiva carenza di medici competenti in diverse Regioni italiane. Quindi, è bene che queste due figure rimangano normate come definito dalle leggi vigenti. Quanto poi all'inserimento del rappresentante dei lavoratori, pare più opportuno che sia inserito nell'ambito degli accordi tra le parti sociali. a cui corrisponderebbe l'abrogazione della lettera *g)*, ho presentato un successivo emendamento che lo riempie di contenuti migliorativi proprio riguardo alle funzioni di queste figure.

626 del 1994. Togliendo la prima parte, l'emendamento risulta indebolito; tuttavia va nella stessa direzione. La Commissione ha approvato una serie di miglioramenti rispetto ai poteri degli RLS, ma credo che essi debbano essere ulteriormente potenziati, e così complessivamente i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici,

sono assolutamente contrario a questo emendamento del relatore, che vuole aggiungere il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Non credo che il contributo del CNEL debba essere disposto in modo così preciso e indicativo in un provvedimento di legge, atteso che esso può comunque

Ricordo che, ad esempio, tra poco esamineremo in Aula - come stiamo facendo in Commissione - la formulazione proposta dal Governo in ordine alla fondazione a cui dev'essere trasferita la proprietà la proprietà della RAI e, quindi, il pacchetto che, in atto, consente al Ministero dell'economia di essere al tavolo...

Credo che questo non sia un sistema giusto; quindi, è giusto reperire i fondi su altri capitoli e non su quello già finalizzato alla riduzione del tasso degli artigiani.

secondo il quale la prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro si deve collegare all'evoluzione della scienza e della tecnica, tuttavia con la previsione di un limite di predeterminabilità oggettivo. il criterio si ispira tanto alla necessità di avere sempre a riferimento, per fortuna, l'evoluzione della scienza e della tecnica con riferimento alla consapevolezza dei rischi per la salute e la sicurezza, ma allo stesso tempo anche assumendo quella certezza del diritto che può essere garantita da un criterio di predeterminabilità oggettiva dell'evoluzione dell'evoluzione stessa della scienza e della tecnica. Abbiamo visto troppo spesso l'intervento di alcune procure con riferimento ad eventi in danno della salute dei lavoratori, ma riferiti a tempi nei quali non era assolutamente predeterminabile il danno connesso ad un determinato materiale o ad un determinato processo di produzione.

più volte all'esame delle Commissioni parlamentari, e torna nella sede opportuna della legge delega per la redazione di un testo unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro. Si tratta di materia che le parti sociali hanno concordato tra loro. Esistono accordi sottoscritti dalle organizzazioni di categoria della CGIL, della CISL e della UIL, e, dall'altro lato, dall'associazione dei costruttori e dalle altre organizzazioni dei datori di lavoro con riferimento a questa intesa, sono state rivolte anche lettere sottoscritte da tutti questi attori al Ministero del lavoro in più occasioni affinché anche questo contenuto delle intese venisse recepito da atti legislativi. Mi riferisco alla esclusione dagli obblighi inerenti il collocamento obbligatorio dei disabili nei cantieri edili e nelle altre attività assimilabili. Qui c'è una evidente contraddizione tra una norma che a suo tempo fu assunta in modo indifferenziato, senza tener conto della specifica caratteristica di un cantiere edile, e condizioni di disabilità fisica o psichica che ovviamente non possono dare luogo ad attività lavorativa in un contesto che metterebbe a rischio l'incolumità di queste persone.

da coloro che non vogliono modificarla; i datori di lavoro la eludono normalmente pagando alla luce del sole la penale che consente di evitare l'assunzione del lavoratore disabile secondo la disciplina del collocamento obbligatorio. Non comprendo la ragione dell'opposizione del Governo, non comprendo l'insensibilità della maggioranza e di quei settori di essa che pure, quando si trovano di fronte alle ragioni della impresa,

perché davvero siamo in presenza di una norma che costituisce rispetto elementare per i disabili e per le ragioni dell'impresa.

permanente di quel fondo di finanziamento degli investimenti rivolti alla promozione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro che già nel passato l'INAIL ha gestito con mezzi trasferitigli dal bilancio dello Stato. Tale esperienza è stata positiva, tutti i Gruppi in Commissione hanno affermato la necessità di prorogare l'esperienza positiva già svolta dall'INAIL, ma il Governo non ha dato la disponibilità

che il fondo sia finanziato annualmente mediante appositi stanziamenti da iscrivere nella legge finanziaria, quindi con un atto di rinvio, ma assumendo qui la ricostituzione del fondo e la decisione che la legge finanziaria ogni anno provveda a finanziarlo.

questo provvedimento è un disegno di legge di delega, quindi dovrebbe rispettare l'articolo 76 della Costituzione. Il Parlamento dunque delega il Governo a legiferare in una materia estremamente complessa e con dei criteri direttivi che mi sembrano talmente vaghi da porsi al di fuori dell'articolo 76 della Costituzione. Tuttavia, su questa parte non possiamo più intervenire, quindi speriamo un intervento dell'altro ramo del Parlamento. L'emendamento 1.36 del senatore Galli prevede che i pareri delle Commissioni competenti sui decreti legislativi che verranno emanati sulla base di questa legge delega

a che i pareri espressi dalle Commissioni competenti - in particolare la Commissione lavoro - non siano vincolanti. Si dà cioè una delega quasi in bianco al Governo dicendogli di fare quello che vuole su tutto il settore della sicurezza e della tutela della salute sul lavoro

il Parlamento si priva anche del potere d'intervenire su svarioni che faccia il Governo in seguito, presentando lo schema del decreto legislativo alla Commissione competente. Rivolgo quindi un appello

allora privare voi stessi della possibilità di esprimere il parere su ciò che il Governo farà con questa delega in bianco? Ma quale ragione c'è? Se voterete a favore dell'emendamento in esame, non vi sarà alcuno sforamento di bilancio, non cadrà - purtroppo! - alcuna maggioranza e alcun Governo; semplicemente resterà in piedi un minimo di possibilità,

anche su questa materia, particolarmente pesanti. Torno a ricordare l'esenzione dai controlli sulla sicurezza del lavoro introdotta dal comma 1198 della legge finanziaria: so che so che non avreste mai votato questa disposizione potendola votare, ma adesso vi si pone la possibilità di dare al Parlamento, alla Commissione, almeno la possibilità di intervenire di fronte agli svarioni, ai mostruosi provvedimenti che eventualmente il Governo dovesse assumere. Volete privarvene? Non eravate voi quelli che, quando si trattava di votare sul *referendum* per la riforma del Parlamento, vi ergevate a vestali, difensori delle prerogative del Parlamento di fare le leggi e vi opponevate ad un Governo che travalica, ad un *premier* dittatore? Era tutta propaganda perché non c'era nulla di tutto questo nella riforma costituzionale. Ora, quando si tratta di agire, demandate e pretendete dal Parlamento che abdichi al proprio potere, lasciando

eserciterà un po' il dovere, stabilito dall'articolo 70 della Costituzione che assegna alle Camere la funzione legislativa.

che però non dà i risultati che il popolo si aspetta. Dunque, per definizione deve essere un intervento di tipo politico. Quindi, ripeto, più giusta sarebbe stata la strada tradizionale di una legge normale; si è scelta la delega e va bene, però, almeno, la possibilità di tenerci qualche giorno di controllo su quello che uscirà dal lavoro del Governo e dei funzionari che lavorano al suo interno, credo che sia il minimo

al di là del significato costituzionale, il fatto che si dia la possibilità - ciò può avvenire quando c'è un Governo di centro-sinistra o di centro-destra - al Governo di ricevere la delega del Parlamento all'emanazione di un provvedimento legislativo e che, poi, questo non sia effettivo e reale, perché il provvedimento legislativo è subordinato al parere vincolante delle Commissioni, esprime una contraddittorietà tra quello che facciamo e ciò che è previsto dall'articolo 76 della Costituzione.

della Costituzione, aveva un significato di modifica della Costituzione stessa e, quindi, soggetto ad altra procedura e non accettabile all'interno di un provvedimento ordinario.

vorrei annunciare il voto favorevole all'emendamento 1.0.16 e anticipo all'emendamento 1.0.17, a mia firma. dei due emendamenti è analogo e in tutti e due i casi l'intenzione dei proponenti è di valorizzare gli organismi bilaterali, cioè quegli organismi che sono promossi dalle organizzazioni rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori di cui il testo del Governo e della Commissione tratta, ma in modo assolutamente insufficiente. Credo sia necessario riconoscere a questi organismi la capacità, anche in termini di sussidiarietà, di sostituire le funzioni pubbliche o comunque di alleggerire e semplificare gli adempimenti che dalle funzioni pubbliche sono richiesti alle imprese. In particolare, nell'emendamento 1.0.17 si ipotizza che nelle aziende sotto i 100 dipendenti, a richiesta dei datori di lavoro, gli organismi bilaterali possano anche effettuare sopralluoghi finalizzati a verificare l'applicazione delle norme vigenti con rilascio di un'attestazione, la quale potrebbe poi dare luogo ad una programmazione delle attività ispettive di vigilanza che consideri prioritariamente attività sottratte al cono di luce delle forme di controllo sociale che si realizzano attraverso gli organismi bilaterali. C'è, purtroppo, e lo devo rilevare, da parte di larghi settori della maggioranza, una diffidenza nei confronti di tutto ciò che può rappresentare cooperazione tra le parti; c'è una sorta di auspicio ricorrente che le parti privilegino il rapporto di tipo conflittuale e ciò in omaggio a ben note ideologie che considerano il lavoro come epicentro più generale del conflitto sociale. Peccato, perché invece quello della salute e della sicurezza è un obiettivo assolutamente si consegue soprattutto nelle imprese diffuse, nell'agricoltura, nel turismo, nell'artigianato, nel commercio, nell'edilizia; si persegue soprattutto attraverso gli organismi bilaterali che rappresentano la cooperazione tra le parti sociali, la loro condivisione di attività di prevenzione, di formazione, di informazione.

Presidente, la mia è una dichiarazione di voto personale che non impegna il Gruppo al quale appartengo. Io non parteciperò al voto sull'emendamento 1.0.204, seppur è un emendamento presentato da me, perché voterei a favore e quindi

in caso di attività nelle quali sono esposti a rischi molto elevati, e di lavoratori che non hanno l'opportuna informazione e formazione professionale. Sì prevede il divieto di utilizzare questi lavoratori, atipici e precari, in mansioni che prevedono appunto rischi elevati, quali il contatto con agenti cancerogeni, chimici, biologici e attrezzature pericolose.

invito i colleghi a valutare con attenzione questo messaggio importante che possiamo dare in riferimento a temi fondamentali e urgenti, quali sono quelli relativi alla lotta alla lotta agli infortuni sul lavoro e ai drammi che si determinano. Si richiede di potere istituire la settimana dedicata alla memoria delle vittime del lavoro.

Settimana dedicata alla memoria delle vittime del lavoro e alla prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro e di vita

ho chiesto di intervenire sul complesso degli emendamenti per avere occasione di interloquire con il Governo. Durante la discussione generale, ho chiesto espressamente al Governo di farci conoscere un elemento che credo avrebbe dovuto fornirci di sua spontanea volontà. Del totale Del totale degli infortuni che si lamentano sul lavoro, quanti sono dovuti a inosservanza delle norme che già esistono e quanti invece sono dovuti a insufficienza delle norme? Quanti infortuni sono avvenuti perché, pur rispettando le norme, queste ultime si sono rivelate insufficienti o è accaduto qualcosa per cui l'infortunio è avvenuto è avvenuto lo stesso? Quanti invece sono classificati come infortuni del lavoro quando nella pratica si tratta di incidenti stradali avvenuti mentre il lavoratore si recava o tornava dal posto di lavoro o si

l'obiettivo è la riduzione degli infortuni sul lavoro, questo è chiaro, ma per capire in quale modo agire, dobbiamo sapere quanti di questi infortuni sono dovuti alla mancata osservanza delle norme che già esistono

sul posto di lavoro), la maggior parte degli incidenti avviene per mancata osservanza delle norme che già esistono, non serve a nulla modificare le norme di sicurezza. Tutt'al più si deve intervenire sui controlli e, forse, sulle sanzioni per la mancata osservanza.

silenzio totale in sede di replica. Quanto meno, per normale rispetto del Parlamento o più banalmente per normale educazione, ad una domanda estremamente pertinente sarebbe gradita una risposta; quanto meno, una spiegazione dell'assenza della stessa. Invece, il Governo nulla ci ha detto in sede di replica; nulla ci ha detto in sede di formulazione dei pareri; nulla ci ha detto in risposta all'interrogazione alla quale, se non seguirà una risposta nel corso della discussione, avrà poco senso darla in seguito, anche se permarrà il mio

se è vero che è qui per sorreggere la maggioranza, è pur sempre Ministro della salute e gli incidenti sul lavoro sono anche competenza sua, quanto meno per capirne le cause; forse dovrebbe anche essere una sua curiosità; forse al telefono sta per l'appunto domandando questa informazione. Ripeto l'appello al Governo affinché risponda alla mia domanda, che non è una curiosità oziosa, ma è fondamentale per capire che cosa stiamo facendo. LEONI *(LNP)*. Anch'io voglio far sentire la mia voce come operatore del settore. Continuo a sentire in Aula situazioni che non mi convincono e diventa anche il mio un appello al Governo a darci delle risposte. risposte. Si fa riferimento continuo alle morti bianche nei cantieri. Sono un operatore del settore e penso che la situazione nasca dalla grande voce del Presidente della Repubblica, che ha preso la parola più volte sulle morti bianche. Allora il Governo corre ai ripari, facendo dei pasticci, però, e ve lo posso anche dimostrare: se le regole

ad un corso, non ha nessuna prova da affrontare. In particolar modo, la sicurezza non la dovete far fare agli architetti o agli operatori di cantiere. La sicurezza viene da lontano e va curata dalla manodopera che opera nei cantieri,

cioè ragazzi che non sono mai stati in un cantiere. I primi a essere pericolosi sono questi ragazzi, che escono dall'università e vanno nei cantieri per fare controlli

precedentemente, che ci fornisce alcune indicazioni che comunque ci permettono di intuire dove accadono gli infortuni più rilevanti. Da questa banca dati, che riguarda in maniera particolare le morti e non ancora gli incidenti che generano infortuni non mortali,

che s'inserisce in quella che prima doveva essere una legge delega e che poi invece aggiunge otto articoli? Ricordo che la legge delega deve essere norma di coordinamento delle leggi esistenti e quindi, di fatto,

che si determinò negli anni 1995, 1996 e seguenti e rispetto a cui oggi probabilmente possiamo osservare una certa regolarità. Vorremmo sentire ancora meglio il relatore e il Governo, per essere sicuri

per una disposizione che arrecherebbe grave nocumento e disarmonia alla legislazione vigente con una difficoltà alla virtuosa intrapresa. Signor Presidente, mi trovo costretto ad intervenire visto che il senatore Ferrara ha evocato gli eventi di quegli anni in maniera forse corretta ma non esaustiva. Ricordo che che fui relatore di questo provvedimento sia sotto il Governo Berlusconi, con il ministro Comino, sia poi con il Governo Dini, con il ministro Treu. fu quello di edulcorare al massimo il testo governativo, perché, lo ricordo, eravamo in presenza di un decreto legislativo e quindi di un provvedimento costruito dal Governo sul quale, come tutti ben sappiamo, il Parlamento non ha non ha possibilità di interventi cogenti ma semplicemente consultivi. Il mio compito di rendere il più possibile accettabile alle aziende il decreto legislativo n. 626 si spinse fino al punto per il quale noi votammo insieme all'opposizione contro la maggioranza; lo devo dire per verità storica, perché anch'io sono convinto (e i dati oggi a dieci anni di distanza ce lo dimostrano) che il decreto n. 626 di fatto ha avuto ben pochi effetti sull'incidentalità del sistema industriale

Come ho già avuto modo di precisare in quest'Aula distratta, non è vero che oggi ci troviamo di fronte ad un'emergenza incidenti, non è vero che ci troviamo di fronte ad un'emergenza mortalità. Certo, il nostro compito e il nostro auspicio devono essere quelli di arrivare a mortalità zero, e ciò è possibile: vi sono aziende estere che hanno ormai da anni all'interno dei propri opifici tassi di mortalità e di incidentalità pari a zero, quindi è un traguardo che è possibile raggiungere.

automatizzati che riducono la possibilità di incidenti, perché l'uomo ormai non lavora quasi più sulla macchina. Dunque, se andiamo a vedere questa curva di discesa ci accorgiamo di un fatto che dovrebbe farci riflettere (anche se non pretendo che quest'Aula rifletta perché è in tutt'altre faccende affaccendata):

in qualsiasi modo, come ho già avuto modo di dire qualche giorno fa, siccome dobbiamo dimostrare di esistere, andiamo a calcare ancora la mano con ulteriori

lavoro. Dal primo giorno, ho inutilmente segnalato - a nome non solo mio, ma di molti altri colleghi - le condizioni di temperatura di quest'Aula. *(Applausi

vi sono correnti d'aria fredda che colpiscono le senatrici ed i senatori, determinando un rischio immanente per la loro salute.

le elezioni in un'unica giornata dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e rafforza il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Si tratta, dunque, di un articolo innovativo che

contrario all'approvazione dell'articolo. Sarebbe stato un voler ripeterci, qualora avessimo fatto una dichiarazione di voto sull'emendamento soppressivo e non sull'articolo finale.

in tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, i programmi di studio delle materie tecnico-scientifiche e giuridiche devono essere riorganizzati in modo che una quota non inferiore al 5 per cento sia dedicata all'informazione e alla formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e alla promozione della cultura della prevenzione. 9. Dalla data di entrata in si parla in modo costante ed insistente di cultura della prevenzione, della cultura della salute nei luoghi del lavoro.

del Governo, che non entra assolutamente nelle competenze del Ministero della pubblica istruzione o addirittura mette in discussione l'autonomia organizzativa ed economica delle scuole e degli istituti:

che più volte e in più circostanze - e le ho potute vivere anche personalmente in dibattiti pubblici - si è sempre espressamente dichiarato favorevole a far sì che la cultura del lavoro, della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro sia quanto più elemento centrale della formazione dei giovani, dei giovanissimi e financo all'università. sottosegretario Patta, la invito a riflettere su questo emendamento, altrimenti andiamo a vanificare i lavori della passata Commissione d'inchiesta che in questo modo si è orientata (mi riferisco alla legislatura precedente), i lavori dell'attuale Commissione d'inchiesta che in questo modo si è orientata (e mi riferisco a questa legislatura), gli orientamenti del Governo, oltre che quelli del Parlamento.

cultura della salute e della prevenzione degli infortuni, affinché fin da bambini si impari ad avere attenzione a questo grande tema.

del Governo. Sono assolutamente convinto del ruolo centrale che ha la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro nei percorsi scolastici; però, c'è una Commissione che sta riscrivendo le indicazioni nazionali dei percorsi scolastici, c'è l'autonomia scolastica ci sono le prerogative proprie del Ministero della pubblica istruzione nel riscrivere le indicazioni nazionali. Credo non si possa imporre in maniera rigida

4. Si ipotizza infatti che i servizi ispettivi possano adottare provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, non solo in presenza di gravi violazioni relative alla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nel lavoro, ma anche - e prego i colleghi di ascoltare con attenzione - nel caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale. e settimanale. Soprattutto nelle aree nelle quali vi è carenza di manodopera è ben noto che, in termini certamente discutibili, tuttavia per ragioni comprensibili, le parti colludono nel ricorrere anche ad un eccesso di straordinari - cosa certamente riprovevole - che, ove rilevata dalle attività ispettive, deve dare luogo a sanzioni. mi sembra assolutamente sproporzionata la sanzione della sospensione dell'attività imprenditoriale per eccesso di straordinario, anche perché si tratta di una misura eccezionale, discutibile anche negli altri casi, perché colpisce i terzi incolpevoli, cioè le lavoratrici e i lavoratori di quella stessa azienda, e interrompe l'attività di impresa che costituisce un interesse generale anche quando le persone che di essa portano la responsabilità abbiano avuto comportamenti in violazione delle norme. delle norme. Pertanto, segnalo all'Aula una particolare attenzione per l'emendamento 4.200, che prevede di sopprimere, almeno limitatamente a questo tipo di violazioni, la sanzione della sospensione dell'attività imprenditoriale per le ragioni che ho ricordato e anche - come ho detto - per la manifesta sproporzione con violazioni relative al lavoro straordinario.

solo dell'argomento del giorno e poi, passato l'interesse specifico per quella tematica, dimenticarsi di tutto e ricominciare a parlare in maniera ideologicamente esattamente opposta.

per il semplice buon senso che in situazioni particolari, se il mercato è quello, si deve agire oppure si perde. Non parlo, poi, di tutti coloro che all'interno della stessa maggioranza di centro-sinistra presentano la Cina come un grande Paese perché la gente lavora sedici ore al giorno e dorme in fabbrica.

è carenza di manodopera specializzata; il mercato è sempre meno prevedibile, per cui vi sono

piedi il Paese, per pagare le tasse, per stare negli studi di settore che voi improvvidamente portate avanti; fanno i miracoli per coprire i buchi che fa Bassolino in Campania e, poi, voi come risultato finale le volete chiudere. Mettiamoci d'accordo allora; se volete veramente salvare il Paese, cominciate a ragionare con un po' di buon senso.

Presidente, vorrei richiamare l'attenzione della maggioranza su certe decisioni di cui poi essa si pente. Per esempio, ieri,

ma in realtà creano il presupposto per un'insorgenza sociale che li potrebbe travolgere storicamente. A quel punto, allora, per la sconfitta elettorale nel Nord, ma per il rischio di un'insorgenza sociale di vastissime proporzioni, hanno deciso di rivedere in parte la politica del Governo. Ora cosa sta avvenendo? Sta avvenendo che questa sinistra profondamente ideologizzata ha imboccato una strada rischiosissima che, come quella degli studi di settore, provocherà delle reazioni, da parte dell'Italia che lavora, che saranno molto dure. Qui c'è una sorta di ideologia dell'interdizione, della sanzione interdittiva. Ci sono dipendenti in nero extracomunitari? Ecco che si decide di interdire l'attività di quella impresa. Ci sono problemi per quanto riguarda gli orari e i tempi di lavoro, il riposo giornaliero e settimanale? Ed ecco la misura interdittiva, si chiude cioè l'azienda. Poi, il terzo incolpevole, cioè il dipendente di quell'azienda, rimane disoccupato e il problema non si pone. Cosa c'è dietro questo tipo di impostazione? Perché si punta alla sanzione interdittiva? Perché, in realtà, la sinistra di classe in questo Paese, che poi è la classe in queste società, interpreta i bisogni del potere bancario, della grande industria e poi dei sindacati operai e delle aristocrazie operaie delle grandi fabbriche. Per questa sinistra di classe, in realtà, la piccola, piccolissima impresa, la microazienda è il nemico giurato; in pratica, verso questo tipo di società si nutre lo stesso odio ideologico dello stalinismo nei confronti dei kulaki.

colleghi della sinistra e del Governo, è quello di rivedere questa impostazione, perché se credete, con questo terrorismo normativo,

i provvedimenti posti in atto per far sì che gli ipermercati spazzassero via la microimpresa commerciale, sta avvenendo invece una ripresa della microimpresa commerciale a scapito degli ipermercati. Infatti, mentre negli ipermercati il livello delle vendite è stazionario, nella microimpresa commerciale l'anno scorso ha subito un incremento del 5,6 per cento. Quindi, in realtà, poi le società si organizzano e si autodifendono. È inutile che seguite la strada di prevenzione e di disincentivazione dell'impresa complessiva diffusa e radicata sul territorio. Ecco perché, cari colleghi, vi invito a riflettere su questo tipo di impostazione, che - guardate - susciterà un allarme sociale tale da provocare un distacco sempre più radicale e forte di quei ceti sociali nei vostri confronti. Stalin distrusse i kulaki deportandoli, provocando una tragedia in quelle parti dell'Unione Sovietica in cui quell'assetto sociale esisteva. Qui Stalin però non c'è, voi siete democratici, siete di sinistra, siete progressisti e allora quelle politiche non le potete attuare. Quindi, alla fine, cosa avverrà? Che sarete sconfitti dai kulaki. Ecco perché, al limite, a noi questo tipo d'impostazione del nostro lavoro legislativo può anche riuscire utile perché alla fine sarete sociologicamente e storicamente sconfitti.

uno degli interventi che veniva ribadito da questa parte politica era che quel provvedimento avrebbe potuto essere riguardato come un semplice emendamento

introdotte con il provvedimento sulla repressione del caporalato avrebbe potuto essere una parte dell'articolo 4 proposto all'approvazione di questa

provvedimento, perché proprio il comma 3 dell'articolo 4 recita: «È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti».

soltanto un significato di bandiera, un significato demagogico, riconosciuto da molti istituti di rappresentanza, imprenditoriali e non, mentre era stato un condizionamento alla politica del Governo e all'espressione di voto di quest'Assemblea da parte della sinistra radicale.

tra persone giuridiche e fisiche o persone che comunque, se non propriamente giuridiche, avevano la gestione di personale in quanto organizzate sotto forma di impresa al momento in cui per quelle organizzate sotto forma di impresa era motivo di inasprimento della sanzione la presenza di un solo lavoratore irregolare, e invece, nel caso in cui il datore di lavoro fosse persona fisica, si poteva prevedere anche la presenza di due lavoratori.

si ha un inasprimento eccessivo a nostro avviso - mi riservo di intervenire sull'emendamento del senatore Poli che propone la soppressione dell'articolo 5 - perché, come diceva poc'anzi il senatore Sacconi, oltre all'inasprimento, che rimane in questo caso costante, e quindi fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, si possono attivare provvedimenti di sospensione dell'attività

in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale. È una situazione che non sta in piedi, signor Presidente, una situazione per cui siamo davvero preoccupati,

è ossessivamente contraria alla libertà di intraprendere, alla libertà di produrre, se non attraverso un lavoro dipendente. Ma che lavoro dipendente potrà esserci se alle imprese non viene data la possibilità

dall'articolo 4, che non tiene conto di una realtà che dovrebbe essere guardata con migliore attenzione, con maggiore prudenza e (signor Presidente, mi permetta, l'ora ce lo consente e i colleghi lo perdoneranno), senza parlare continuamente al telefono così come fa il rappresentante del Governo, così come fa il Ministro della salute, non già dimostrando una scarsa sensibilità o attenzione a quello che diciamo forse impropriamente o con un modo di vedere assolutamente diverso dal loro, ma con un dileggio delle istituzioni che non tiene conto di quello che un lavoro parlamentare dovrebbe consentire, cioè il confronto e non già, a questo punto, la disattenzione totale.

esprimerà parere favorevole avendolo scritto lui, assegna gli stessi poteri anche alle aziende sanitarie locali

A parte il testo costituzionale, dovrebbe essere ben chiaro a tutti (forse questo andrebbe chiarito nelle scuole assieme alle mille cose che si vuole che nelle scuole si insegni) che tutto quello che noi abbiamo, tutto ciò che costituisce una risorsa

anche una sospensione provvisoria, può voler dire un colpo mortale per questa attività imprenditoriale che, secondo l'articolo 41 della Costituzione, è libera.

Infatti possiamo immaginare che il lavoratore venga pagato ugualmente anche se c'è un fermo imprenditoriale, ma può essere un fatto del tutto transitorio; in alcuni casi, un fatto talmente transitorio da non poter sussistere, perché evidentemente un'azienda che è in queste condizioni può facilmente arrivare alla Allora, siamo sicuri che sia sensato attribuire poteri così ampi agli ispettori del Ministero del lavoro e al personale dell'azienda sanitaria locale, laddove le garanzie che generalmente vengono richieste per atti assai meno rilevanti assolutamente non ci sono? sono? Noi rischiamo di dare un colpo mortale ad aziende e consegnare questo potere non a magistrati - che, quantomeno, devono conoscere certe procedure legali - ma a persone che hanno competenza di un altro tipo:

credo che questo articolo sia di particolare importanza. Vorrei innanzitutto sottolineare che non siamo animati dalla volontà di perseguire le imprese;

rivolta anche su una materia come questa al sistema delle piccole e piccolissime imprese, vitale per il Paese

agli anni '60 e '70, sono in calo. Tuttavia - la cronaca di tutti i giorni lo rimarca - ahinoi! - siamo in presenza di numeri, anche a metà di quest'anno, davvero gravi ed allarmanti. Non siamo ancora al completamento del del semestre e gli infortuni mortali sono già arrivati a 500! È una piaga sociale che deve essere affrontata - insisto - anche con provvedimenti legislativi, che non vogliono - ripeto colpire le imprese, ma tutelare il lavoro e garantire alle imprese una prestazione lavorativa sicura, la soluzione migliore per mettere le imprese in quelle condizioni di produttività che spesso non ci sono. L'articolo, in particolare, affronta affronta due argomenti: il primo riguarda il coordinamento necessario delle attività di vigilanza e di prevenzione. Si è detto anche nella 11a Commissione - ed emerge ciò anche

Anche questa non è un'indicazione casuale: pensiamo che sia soprattutto il livello territoriale che va attivato per svolgere un'attività di vigilanza, che - insisto - soprattutto a questo livello, dev'essere coordinata, oltre che naturalmente

violazioni delle normative della sicurezza. Ci sembra utile - per venire all'emendamento 4.800 che ho riformulato - che questo potere venga dato anche alle ASL e non solo agli ispettori, per le ragioni che prima cercavo di evidenziare: cioè, la prevenzione e anche una più efficace attività di vigilanza si può esercitare soprattutto a livello territoriale, utilizzando tutte le risorse disponibili. FERRARA

che ho presentato con carattere di urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento. Debbo dire che, con solerzia apprezzabile, il ministro Di Pietro, uno dei tre destinatari, mi ha risposto il giorno dopo con una sua missiva, dicendomi che si sarebbe occupato dell'oggetto dell'interrogazione. Essa riguarda situazioni scabrose che si verificano sulla testata della pista dell'aeroporto di Ciampino,

È vero, oggi non abbiamo parlato, ma durante la scorsa legislatura abbiamo rivendicato il diritto dei familiari delle vittime ad essere risarciti e a conoscere la verità ed i colpevoli. Per anni il Governo di centro-destra non ha fatto nulla. Il senatore Ferrara dimentica che le aspettative dei familiari e i lunghi anni di attesa hanno avuto un riscontro nella finanziaria dello scorso anno. Nei fatti, l'attuale maggioranza ha dato una risposta concreta: i familiari hanno diritto al risarcimento perché i morti di Ustica vengono considerati come vittime del terrorismo. Ricordo che quella finanziaria fu votata dall'Unione con i voti contrari del senatore Ferrara e di tutta la Casa delle Libertà.

un mio intervento reso in apertura di seduta che non aveva soltanto il significato di richiamare alla memoria la strage di Ustica, ma puntava a stigmatizzare il comportamento della maggioranza

non perché da parte nostra ci sia un atteggiamento dilatorio e ostruzionistico, ma perché vi è inefficienza e scarsa capacità